anni or sono, il 1° dicembre 1999, scompariva Luigi Granelli, per diverse legislature membro autorevole di questa Assemblea e Vice Presidente del Senato dal 1992 al 1994. Nato a Lovere, in provincia di Bergamo, nel 1929, cominciò sin dalla giovinezza ad affiancare alla sua attività di operaio tornitore un fecondo cammino personale di formazione culturale e spirituale. I suoi studi lo condussero allora a confrontarsi con i più avanzati contributi filosofici e politici elaborati in seno al cattolicesimo francese, dall'umanesimo integrale di Jacques Maritain al personalismo cristiano di Emmanuel Mounier. Lo sviluppo di una concezione esigente del rapporto tra fede cristiana ed impegno politico - nella quale la prima è fonte di valori ed il secondo costituisce lo strumento per l'assunzione diretta delle responsabilità civili e sociali del cristiano animò allora la scelta di Luigi Granelli di militare, fin dai primordi della sua fondazione, per il partito della Democrazia Cristiana, e successivamente, nel 1953, lo condusse a partecipare alla costituzione del movimento della "Base", all'interno del partito. Fu eletto deputato, per la prima volta, nel 1968, nelle liste della Democrazia Cristiana, e rieletto nel 1972 e nel 1976. Nel 1979, al principio della VII legislatura, entrò per la prima volta a far parte della nostra Assemblea, nella quale fu confermato dal corpo elettorale in tutte le successive legislature fino alla XI, nella quale svolse inoltre - come ho già ricordato - le delicate ed autorevoli funzioni di Vice Presidente del Senato. Fu Sottosegretario di Stato per gli affari esteri dal 1973 al 1976, ed in questa veste si occupò in particolare dell'emigrazione italiana nel mondo, organizzando, nel 1975, la prima Conferenza nazionale dell'emigrazione. Dal 1983 al 1987 fu Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica nel primo e nel secondo Governo Craxi e nel sesto Governo Fanfani. Alcune sue iniziative di quella stagione, dalla costituzione dell'Agenzia spaziale italiana alla fondazione a Trieste del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, diedero diedero un chiaro segnale di attenzione, da parte delle istituzioni, verso i problemi della ricerca, e contribuirono ad una prima inversione di tendenza di quella vera e propria diaspora dei nostri migliori ricercatori che, in quegli anni, rischiava di minare le prospettive di sviluppo del nostro Paese. Dal 1987 al 1988 fu infine Ministro delle partecipazioni statali nel Governo Goria. A partire dal 1994, deciso a favorire il rinnovamento, anche generazionale, della funzione rappresentativa, scelse di rinunciare alla candidatura al Parlamento; continuò però a porre la sua esperienza e la sua passione politica al servizio del dibattito interno e dell'azione del partito per il quale militava. Fino all'ultimo, nonostante la grave malattia che lo aveva colpito, non cessò di partecipare - con l'acume ed il rigore che gli erano riconosciuti da tutti, amici ed avversari - alle vicende politiche del Partito Popolare Italiano. In uno dei suoi ultimi interventi pubblici, pochi giorni prima della sua scomparsa, Luigi Granelli sviluppò un'accorata riflessione sui destini del cattolicesimo democratico all'interno del sistema politico italiano. Alcuni passaggi di quel discorso, che ammonivano sui rischi che si corrono in ogni istituzione quando all'interno scompare il dibattito sulle idee, costituiscono ancora, a dieci anni di distanza e in un contesto politico assai differente, un prezioso stimolo alla riflessione per tutti noi. Sono certo allora di esprimere la volontà di tutta l'Assemblea nell'esprimere, nel ricordo commosso di Luigi Granelli, un affettuoso saluto alla sua famiglia ed a quanti sostennero, con il loro voto, la sua lunga e feconda attività all'interno delle nostre istituzioni.

sento il dovere di intervenire, avendo avuto con l'onorevole Granelli la stessa militanza e la stessa esperienza nella Democrazia Cristiana e nel Partito Popolare.

sono stati ricordati anche in quest'Aula (Mattei, Marcora, Galloni, De Mita, Bianco), credo che la scuola milanese abbia condotto una battaglia all'interno del partito dei cristiani

Questa scuola gli è servita per inaugurare negli anni Sessanta, anche contro il volere di certa gerarchia ecclesiastica, l'alleanza con il Partito socialista;

nel nuovo Stato, il rapporto che i cattolici hanno avuto con i liberali e con i marxisti, esprimendosi in modo particolare nel periodo dell'unità

avvenuta dopo un discorso fatto al congresso di Rimini del Partito Popolare, è emblematica ed indicativa. Non possiamo che ricordare

È stato sempre parte di una minoranza, ma di una minoranza scomoda. Credo che qualche suo insegnamento serva anche oggi. L'insegnamento che ho tratto dai suoi scritti (è stato anche un pubblicista molto prolifico)

La sua vita e la sua storia possono essere un esempio per tutti noi, per l'impegno e la passione posti nello svolgere l'attività politica. L'ambiente in cui Granelli matura le proprie convinzioni ed opera le prime scelte di campo ideologico e politico è quello del mondo del lavoro e della gioventù di Azione cattolica. Queste due esperienze segneranno il suo percorso politico, che lo porterà ad avere un approccio laico alla politica pur essendo un uomo di fede. Partecipò sin da giovanissimo alla Base, corrente DC che affermava l'autonomia politica dei cattolici combatteva i tentativi di apertura a destra delle maggioranze parlamentari, lanciando proposte riformiste in materia economica, sociale ed istituzionale. La sua anima critica lo rese un personaggio scomodo sia all'interno che all'esterno della DC, ma ricevette sempre la stima sia dei suoi colleghi di partito che degli avversari politici, stima dovuta soprattutto al suo impegno politico e alla sua coerenza. Granelli è stato protagonista di una carriera politica di assoluto livello; si spese sempre al massimo in ogni incarico cercando sempre di lavorare in funzione del bene comune e per lo sviluppo di questo Paese.

Le posizioni del cattolicesimo democratico e della sinistra italiana sono state sempre alla base del suo impegno politico. Onorevoli colleghi, Granelli ci ha insegnato che la politica non è fatta di interventi astratti e di trasformismo, ma piuttosto di coerenza e di politiche condivise e giuste per il Paese.

una delle principali personalità della storia della nostra Repubblica, figura emblematica del cattolicesimo politico, di cui per oltre mezzo secolo è stato un animo irrequieto. Per chi, come me, da giovane, insieme a tanti altri, si è avvicinato alla politica seguendo le idee e l'azione del compianto Vice Presidente del Senato, l'emozione in quest'Aula è davvero forte.

operaio all'Italsider, uomo di Governo, sincero democratico, coerente pacifista, impegnato in tante giuste battaglie per combattere le disuguaglianze e i disagi umani e sociali del Paese. Uomo della Democrazia Cristiana, intimamente legato a Marcora, con un gruppo di militanti in larga parte giovani, a Belgirate, sul lago Maggiore, contribuì alla fondazione della Sinistra di Base, per dare un nuovo respiro all'iniziativa delle forze di sinistra nel partito di ispirazione cristiana. I valori di giustizia sociale, di promozione e affermazione dei diritti del lavoro, a cui ha ispirato tutta la sua partecipazione politica, nascono dall'esperienza giovanile in fabbrica, dove entra in contatto con quei gruppi sindacali e politici che considerano questi quali essenziali valori democratici. La partecipazione all'Azione Cattolica gli permette di entrare in contatto con le principali espressioni del cattolicesimo europeo - Maritain e Mounier elaborando così le sue teorie sullo sviluppo della società e sui rapporti tra fede e politica. Non possiamo che emozionarci ricordando un uomo che nella sua esperienza politica ha affrontato, con posizioni oltranziste, temi oggi attualissimi. Fu Granelli, infatti, come uomo di Governo, da sottosegretario per gli affari esteri, ad interrompere il tradizionale disinteresse della politica nazionale verso i nostri emigrati all'estero, come lei ha già ricordato, Presidente. Fu Granelli, come Ministro della ricerca scientifica, ad aumentare con decisione la spesa per la ricerca, a istituire un laboratorio per le biotecnologie a Trieste, a costituire l'Agenzia spaziale italiana, ad autorizzare l'insediamento della macchina di sincrotrone affidandolo alla guida del premio Nobel Rubbia per contrastare la fuga di cervelli, consapevole dei danni che questa aveva e avrebbe causato impoverendo per decenni il mondo della ricerca scientifica nazionale. Fu sempre Granelli, pur essendo all'epoca Ministro delle partecipazioni statali, a promuovere la privatizzazione di Mediobanca e della Lanerossi, ma a opporsi fermamente all'accordo ENI-Gardini sul progetto Enimont intuendone i termini che avrebbero causato la crisi e il fallimento. Durante i suoi mandati parlamentari spesso assunse posizioni diverse rispetto a quelle ufficiali della DC, ma sempre facendo valere la propria autonomia di giudizio e la propria obiezione di coscienza limitatamente alla fase di contributo al dibattito per la definizione dei provvedimenti, rientrando sempre nei limiti della disciplina del partito nelle fasi conclusive del voto. Meritano a questo proposito di essere ricordate, su tutte, le sue battaglie contro la legge Mammì sull'emittenza radiotelevisiva, frutto della perspicace intuizione riguardo la condizione di privilegio che si andava delineando. Oggi, ancora una volta, è giusto rendergli omaggio per l'intensità della sua partecipazione alla battaglia delle idee, per la sua costante presenza in ogni fase del dibattito politico, per l'impegno affinché venissero assicurati i rapporti di forza nella società e nelle istituzioni. Granelli, maestro e discepolo del pensiero democratico e cristiano, interprete autentico del cattolicesimo politico, uomo del Novecento, mite e generoso, sempre pronto a combattere sulle barricate delle cose difficili, laico nella sua fede, profetico nel suo agire, ha saputo cogliere fino in fondo lo spirito profondo che emerge dal messaggio del bresciano Cardinal Bevilacqua, laddove nel 1925 davanti ai fascisti che volevano soffocare la sua limpida voce di libertà e minacciavano di fargli pagar care le sue idee, rispondeva «Le idee non valgono per quello che rendono, ma per quello che costano». Granelli, cari amici, ha vissuto cosi, rifiutando ogni rassegnazione in un tempo fortemente carico di incertezze, con quell'animo limpido e cristallino che consegna a noi, colleghi senatori, a quest'Aula, alle future generazioni, il senso pieno della memoria di futuro. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord si unisce con rispetto al ricordo di Luigi Granelli a dieci anni dalla sua scomparsa. Lo ricordiamo - è già stato detto da altri parlamentare per tante legislature, espressione di quei cattolici democratici impegnati in politica che trovarono nella Democrazia Cristiana la casa e lo strumento per la loro militanza. In particolare, Luigi Granelli frequentava molto spesso Lecco - la mia città - e la sua provincia per i legami con quella Sinistra di Base democristiana che aveva in Albertino Marcora il suo leader. Ho citato Albertino Marcora proprio per riandare ai tempi della Resistenza partigiana, che vide appunto Marcora e Granelli impegnati insieme, sia pure su fronti diversi. Non a caso, il richiamo ai valori antifascisti fu la costante della vita e dell'azione politica di Granelli; un personaggio, una coscienza critica che a volte tornava scomoda ai suoi stessi amici. l'impegno fu totale per una Repubblica democratica fondata sulle autonomie. Non a caso il regionalista don Luigi Sturzo fu uno dei suoi punti di riferimento. Rivestì con rigore e coerenza cariche di partito e di Governo, con quello spirito di servizio che anche gli avversari gli riconoscevano, perché Granelli era un politico lontano dagli interessi particolari e personali, ma sapeva stare tra la gente per coglierne le esigenze concrete e ideali.

è già stato detto, ma, con emozione, mi soffermerò su qualche passo saliente che dà il senso dell'attualità del ricordo di Luigi Granelli. Luigi Granelli era stato operaio alle acciaierie Italsider e, con un pizzico di civetteria, ricordava sempre questa esperienza come fondativa e qualificante. Soprattutto quando fu Ministro della ricerca scientifica e Ministro delle partecipazioni statali ebbe modo di dimostrare quanto la sua esperienza di lavoro, unita alla sua scelta politica, collocava la dimensione nazionale (ma non nazionalista) del suo impegno per un'Italia che sapesse far tesoro delle capacità lavorative, giocando i suoi talenti in positivo, mettendo le risorse di tutti al servizio di tutta la Nazione, dando un ruolo fondamentale in questo alla dimensione umana e comunitaria del lavoro. Nel senso del bene comune, le partecipazioni statali giocavano in Granelli un ruolo di guida, di avanguardia, di interpretazione al passo con i tempi, delle necessità di ammodernamento del sistema industriale italiano. I lavoratori, come i ricercatori, come i manager, non erano semplici numeri o pedine, ma protagonisti del lavoro creando dignità e condivisione. Luigi Granelli, nato, vissuto e tornato a morire nel suo paese di Lovere, in provincia di Bergamo, fu certo uomo del Nord, uomo che ci fece amare il Nord d'Italia, come luogo non solo dei record produttivi, ma come Nord capace di comprendere e lottare per ridurre le disuguaglianze del Sud d'Italia e del mondo. La sua visione era quella di chi, partendo dal suo territorio, sapeva collocarlo nel mondo. Il suo essere Nord era internazionale, aperto alla scoperta delle contraddizioni della disuguaglianza, volto a proporre metodi comuni di lotta alle clientele, al familismo, alla non integrazione; ci convinceva e ci faceva sognare l'Italia unita, un'Europa federale e solidale, un mondo di fraternità possibile. Era un uomo del Nord con una profonda visione internazionalista, con lo spirito libero ed ironico di un Bertoldo. un Bertoldo. Questa visione internazionalistica Granelli ebbe modo di dispiegarla nel suo impegno politico nella Commissione esteri del Senato e come Vice Presidente di Palazzo Madama. Studiò, elaborò, propose. Ed agì. Quando fu Sottosegretario agli esteri negli anni 1976-1979 egli, nel fuoco delle vicende internazionali delle nascenti (e purtroppo ricorrenti) dittature del Sudamerica, fu, a nome dell'Italia tutta, il promotore istituzionale della posizione ferma e irrevocabile del nostro Paese per la democrazia. In special modo, nei giorni e nei mesi della dittatura argentina, decise l'apertura piena della nostra ambasciata a uomini e donne che scamparono la triste sorte delle migliaia di *desaparecidos*. Noi abbiamo l'onore e la fortuna di avere nel nostro consesso una collega che lottò contro quella dittatura argentina, la senatrice Mirella Giai *(Applausi della senatrice Negri)*. Lei, meglio di me, potrebbe dirvi cosa rappresentò per migliaia di famiglie, moltissime di origine italiana, sapere che le nostre ambasciate e il nostro Governo erano risolutamente contro le brutali dittature sudamericane. Fatti, non parole, quelli di Granelli. Uno stile, quello di Luigi Granelli, che non conosceva sconti per la propria parte politica sui temi dei diritti umani. Sui fatti del Kosovo non esitò a criticare il debole ruolo del nostro Paese e del Governo «amico» quando si decise una serie di bombardamenti a cui l'Italia prese parte prima ancora di informare le Camere, come prevede invece, non a caso, la nostra Carta costituzionale. La vera lotta per la pace per Luigi Granelli era la vittoria del diritto e della ragione, non la scorciatoia delle visioni unilaterali. Questo introduce il Granelli democratico cristiano, meglio ancora cattolico democratico intransigente, che, come ebbe a spiegare più volte, non vuol dire incapace dell'uso flessibile della politica. Dopo tutti gli anni nella DC, fu tra coloro che non volevano cambiare nome alla DC per passare al Partito Popolare. Non vi era contraddizione in un uomo di partito e anche di Governo. Semplicemente non accettava l'idea - lo disse in organi politici della DC e in interviste - che nella notte tutte le vacche potessero essere considerate nere. Colleghi, si è detto la scorsa settimana che il comportamento onorevole - e lo è di molti della DC, e non solo, fu di accettare il giudizio quando toccò loro. La verità è che Granelli, come moltissimi nel suo partito, non dovette mai gridare in un comizio alle Camere che le sue mani erano pulite, perché le sue mani erano davvero pulite. la questione riguardi solo gli iscritti ad un partito, ma, poiché ognuno deve far conto per la propria parte, voglio ricordare che Granelli s'inserisce in un filone che da Murri a Sturzo a Dossetti a Zaccagnini, passando per tanti esponenti del cattolicesimo democratico, era teso anche al rinnovamento della Chiesa, quanto mai necessario in quest'epoca di appannamento del Concilio Vaticano II. Testimoniare, per Granelli, significa testimoniare una tradizione che non muore, che vuole essere di tutti e non di parte, che si vuole fare lievito nella società. Concludo, signor Presidente, ringraziando la Presidenza del mio Gruppo e il Senato per il privilegio concessomi di ricordare Luigi Granelli, che mi avrebbe redarguito per la retorica necessariamente insita ma poi, forse, con il suo splendido sorriso di sempre, mi avrebbe perdonato per la testimonianza di affetto e di verità per lui, ma soprattutto di amore e passione per la politica, che egli ci ha insegnato e di cui speriamo di essere degni. Grazie, Luigi! Grazie,

Ex operaio, partecipò all'Azione Cattolica, fu militante e dirigente della Democrazia Cristiana e successivamente del Partito Popolare Italiano, dal quale alla fine si allontanò. Propugnatore del dialogo con tutte le forze democratiche, fu deputato; ricoprì la carica di Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri durante i Governi Rumor e Moro. Fu membro del Parlamento europeo (con funzioni di capo delegazione della DC), dal 1976 al 1979. Fu anche senatore della Repubblica. Negli anni Ottanta, fu Ministro della ricerca scientifica e tecnologica durante i Governi Craxi e Fanfani e Ministro delle partecipazioni statali durante il Governo Goria. Dal 1992 al 1994 fu Vice Presidente del Senato. La sua carriera parlamentare si concluse per scelta, non perché non fosse cercato e richiesto: smise per permettere alle nuove generazioni di potersi affermare. Questa è, succintamente, la scheda di Luigi Granelli, che fu figura di rilievo nella vita politica e culturale del Paese e che per le idee e i progetti che promosse continua a essere un politico attuale, un uomo dei nostri giorni. Un politico che aveva a cuore il Paese, la società, le persone, i valori da infondere ai giovani, la possibilità di innovare in Italia, di creare occupazione, di migliorare la *performance* della pubblica amministrazione, di essere concreti - più fatti meno parole - di evitare uno sviluppo industriale irrazionale, di favorire una cultura della legalità quale condizione essenziale per la democrazia, di opporsi a chi, anche all'interno della DC, era fanatico nel volere la fine della DC stessa e nell'usare gli avvisi di garanzia per fare posto a una nuova nomenclatura. Negli anni Ottanta, nel settore delle nuove tecnologie e delle scienze applicate offrì supporto e inaugurò il laboratorio SGS ad Agrate, in Brianza,

CARRARA *(PdL)*. Un approccio prima ancora che politico di visione delle cose, pensando a ciò che quello specifico settore dell'innovazione scientifica e tecnologica avrebbe potuto ricevere da quell'area della Lombardia vicino a Milano, ma anche a tutto quello che poteva generarsi in quell'area: un'industria che esige, per affermarsi e crescere, una rete di conoscenze e di relazioni con le università, con altre imprese, con centri di ricerca, con gli Enti locali e la Regione, un tessuto complesso che si crea nel tempo e che porta al consolidamento di un sistema di imprese che determina un *assett* importantissimo per il territorio. Sostenne quindi, con il suo primo direttore, il premio Nobel Abdus Salam, il rafforzamento del Centro internazionale di fisica teorica (ICTP), di Trieste, voluto dall'UNESCO;

promosse la legge su Eureka; nel settore dell'economia e dell'impresa, favorì la privatizzazione di Lanerossi (allora facente parte del Gruppo Eni) e di Mediobanca, cioè l'approvazione da parte del Governo del piano che metteva in perfetta parità il capitale pubblico e quello privato di quest'ultima. Sostenne con partecipazione sentita l'influenza positiva che l'innovazione tecnologica poteva avere sul sistema produttivo, sui processi di modernizzazione, sulla capacità dei servizi di rispondere alla domanda sociale, sull'organizzazione del territorio. Chiuderei questo ricordo del nostro collega e mio conterraneo con alcune sue parole, per far comprendere quanto fosse calato nella storia, nella vita del Paese, quanto ci tenesse a migliorare l'Italia e renderla moderna: "Ci sono uomini come Mattei, Kennedy, Martin Luther King, Moro, dotati di un profondo senso della storia che hanno riempito un'epoca e che sono stati assassinati per le loro idee,

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 17 dicembre. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi è integrato con l'inserimento al primo punto delle ratifiche di accordi internazionali già all'ordine del giorno di giovedì scorso. Seguirà la discussione del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali. Resta confermato che domani, alle ore 16,30, saranno discusse le mozioni sulle riforme costituzionali per le quali i tempi sono stati ampliati fino a 30 minuti per ciascun Gruppo. Sempre nel corso della settimana corrente saranno posti all'ordine del giorno, ai soli fini - come concordato tra i Gruppi - del rinvio in Commissione per un ulteriore approfondimento, i disegni di legge sul reato di tortura fatti propri dal Gruppo del Partito Democratico. Sarà inoltre discussa la mozione Baio ed altri sui malati di diabete. La prossima settimana, nelle sedute del 9 e 10 dicembre, il calendario prevede la discussione di mozioni su temi di ampia condivisione in materia di italiani all'estero, partecipazione dell'Italia alla Convenzione sull'aiuto alimentare e persecuzione dei cristiani, con particolare riguardo all'Africa, nonché di eventuali altre mozioni concordate tra i Gruppi. Nelle sedute dal 15 al 17 dicembre saranno discussi i disegni di legge relativi alla riforma della contabilità e finanza pubblica e alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché il decreto-legge sui concorsi per dirigenti scolastici - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - e ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Nel corso di tale settimana potrà inoltre essere esaminato il disegno di legge sulle cure palliative, se concluso dalla Commissione.

*relatore*. Signora Presidente, il provvedimento, che è già stato approvato da noi in prima lettura, ha subito alla Camera dei deputati alcune modifiche molto limitate, sulle quali dobbiamo esprimerci. Se me lo consente, allegherei mia relazione, nel quale do atto alle modifiche apportate alla Camera di aver ampliato il raggio di verifica parlamentare

Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per manifestare una sostanziale posizione di accordo sul provvedimento in esame da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori. Già nella prima lettura, l'Italia dei Valori aveva manifestato il proprio favore alla ratifica dell'accordo, in quanto, nonostante vi fossero alcune perplessità sull'eccessiva ampiezza della delega conferita al Governo e sui provvedimenti attuativi, riconosceva la necessità di tutelare quanto prima i diritti degli operatori del settore e dei creditori in genere. Il lavoro della Camera in questo senso è stato proficuo, e posso dire che il nostro bicameralismo perfetto, spesso criticato, in questo caso, come in quello del disegno di legge n. 1500, ha permesso che nel passaggio dal primo testo al testo B si operassero quelle modifiche che l'Italia dei Valori aveva proposto. Alla Camera dei deputati, infatti, in accoglimento del parere espresso dal Comitato per la legislazione, si è introdotto un ulteriore comma 3 all'articolo 3, per cui gli schemi dei decreti legislativi ivi previsti sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

il ruolo dell'Assemblea parlamentare rispetto alla gestione di politica estera di esclusiva competenza del Governo, come purtroppo appare in questa legislatura, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori sul disegno di legge n. 1754-B di ratifica dell'accordo in

sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. Art. 2.

alle raccomandazioni di organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. L'attuazione di questo Accordo favorirà l'incremento del flusso di investimenti italiani nella Repubblica

Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anche qui brevemente per manifestare il favore del Gruppo dell'Italia dei Valori sul provvedimento in esame. Come già descritto dal relatore del provvedimento, si tratta della ratifica di un accordo tra il nostro Paese e il Governo della Repubblica di Panama volto a promuovere gli investimenti nei due Paesi, soprattutto tramite la protezione degli stessi attraverso strumenti giuridici riconosciuti e promossi anche da organizzazioni internazionali. Nel caso di specie, non mi soffermerò sulla disamina dell'articolato che compone l'Accordo, ma, fatte salve le riserve già sottolineate durante l'esame in Commissione dal collega Perduca sul comma 4 dell'articolo 10 dell'Accordo, riguardante le procedure di arbitrato, vorrei sottolineare la tempestività con la quale il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica in questione e la celerità con la quale questo ramo del Parlamento lo ha discusso ed oggi sicuramente lo licenzierà. Come tutti in quest'Aula sanno, siamo abituati a tempi a dir poco biblici per la ratifica di accordi particolarmente importanti sia per il nostro Paese che magari per la salute e i diritti di miliardi di persone nel mondo: penso alla cooperazione allo sviluppo, ai protocolli di messa al bando di alcuni armamenti, alla protezione dell'ambiente. Siamo così tanto abituati a questi tempi che non ci può non stupire il fatto che in sette-otto mesi mesi si sigli un Accordo a livello di diplomazia e che questo sia anche approvato dal Parlamento. Come si suol dire, a pensar male non si fa peccato, ma diciamo che degli interessi urgenti di qualcuno a Panama potrà giovarsi anche qualcun altro (o molti altri), soprattutto in termini di aumento dei servizi e della qualità della vita della popolazione panamense e non di pochi eletti. Per questi motivi il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà favorevolmente su questo provvedimento. **Saluto

avremmo dovuto ratificare tutta una serie di trattati internazionali, approvazioni che poi slittarono perché i tempi non lo consentirono.

chiedo il voto elettronico su questo provvedimento, perché ritengo che debba rimanere agli atti, in particolare, la presenza dei membri del Gruppo del Popolo della Libertà, non soltanto continuano a consegnare le loro relazioni, non facendo quindi conoscere nel merito i provvedimenti al nostro esame, ma neanche partecipano, sia come relatori sia anche come votatori, a questo esercizio che, in effetti, ci sta facendo diventare la legislatura maggiormente prolifica. Chiedo

l'accesso al mercato interno dell'Unione europea, ad esclusione dei settori di agricoltura e pesca. L'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede, altresì, una più stretta collaborazione fra le parti nei settori di ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente, politiche sociali, statistica, turismo, diritto societario e protezione dei consumatori. Ogni Paese europeo che aderisca all'Unione europea può chiedere di divenire parte contraente anche dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Occorrerà, quindi, un accordo tra il richiedente e i tre Paesi che che compongono l'Accordo sullo Spazio economico europeo. Con l'adesione all'Unione europea che, come è noto, è decorsa dal primo gennaio 2007, anche la Bulgaria e la Romania hanno chiesto di entrare a far parte dell'Accordo SEE ed è stato raggiunto l'Accordo che è oggetto della presente ratifica (oltre a specifiche intese bilaterali con Norvegia e Islanda). Con l'accesso di Romania e Bulgaria,

Islanda, Liechtenstein e Norvegia), per un totale di 500 milioni di consumatori. I negoziati hanno subito un prolungamento dovuto alla difficoltà di trovare un'intesa sui contributi finanziari che i Paesi EFTA/SEE si sarebbero dovuti impegnare a versare per lo sviluppo regionale di Bulgaria e Romania e le collegate concessioni in favore di Norvegia ed Islanda nel settore della pesca (il Liechtenstein, come è noto, alla pesca non è interessato). l'Accordo consta di sette articoli e due allegati e definisce i necessari adempimenti che verranno recepiti nel testo dell'Accordo SEE, a livello di adattamenti tecnici e periodi transitori, provenienti per lo più dal Trattato di adesione. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che Bulgaria e Romania diventino parti contraenti dell'Accordo SEE e l'articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie al testo principale dell'Accordo e ai relativi Protocolli. L'articolo 3 coordina i mutamenti indotti dalle nuove adesioni agli atti richiamati nell'Accordo SEE. L'articolo 4 stabilisce l'inserimento delle disposizioni elencate nell'allegato B. L'articolo 5 regola le controversie sull'interpretazione o l'applicazione. L'articolo 6 dispone la ratifica dell'Accordo secondo le rispettive procedure nazionali. L'articolo 7 concerne il regime linguistico. L'Accordo è corredato di due allegati. L'Allegato A indica gli atti di cui all'Accordo SEE modificati dall'Atto o dal Protocollo di adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea; l'Allegato B contiene le misure transitorie applicate ai due Paesi per l'attuazione dell'*acquis* comunitario relativo al mercato interno. Gli Accordi e i Protocolli riguardanti le intese intercorse fra Islanda e Norvegia e l'UE e richiamati nell'articolo 6 dell'Accordo non sono stati incorporati nell'Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi dell'Unione europea. All'accordo principale sono allegate alcune dichiarazioni, rese da una, più o tutte le parti contraenti, riportate nel testo dell'Atto finale. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, propongo l'approvazione del

per l'entrata in vigore definitiva di questo strumento è necessario che tutti gli Stati membri, compresa l'Italia, completino le proprie procedure interne di ratifica dell'Accordo. L'estensione ai nuovi membri dell'Unione europea delle disposizioni previste dall'Accordo in tema di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dei capitali promuoverà un ulteriore accrescimento del volume degli scambi, con ripercussioni favorevoli per gli operatori economici europei, in particolare quelli italiani che, come è noto, sono particolarmente attivi in Bulgaria e soprattutto in Romania. Il completamento dell'*iter* di ratifica dell'Accordo in questione costituisce, in sintesi, una condizione necessaria per completare l'adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania,

Come affermato dal relatore, questo Accordo disciplina la partecipazione della Romania all'Accordo sullo Spazio economico europeo il quale vige fin dal 1994 non solo tra i Paesi membri dell'Unione europea, ma anche fra quelli extracomunitari che appartengono all'EFTA (Islanda, Norvegia). La finalità dello Spazio economico europeo è quella di allargare la collaborazione economica Colleghi, per cortesia.

è quella di allargare la collaborazione economica con Paesi non membri dell'UE, rendendoli parte del mercato unico che costituisce la forza dell'Europa nel mondo e lasciando tuttavia esclusi alcuni settori particolarmente sensibili e forse ancora sottostanti a logiche nazionali, come l'agricoltura e la pesca. La Romania e la Bulgaria fanno parte dell'Europa fin dal 2007, ed è quindi fondamentale che le stesse diventino parte integrante anche del SEE, poiché solo con una completa partecipazione a tutte le politiche e le cooperazioni di marchio comunitario si può avere una reale europeizzazione dei Paesi nuovi membri. Lo dico francamente, cari colleghi: io credo poco all'Europa a due velocità, cui alcuni Stati registrano forme di cooperazione più stretta di altri, perché mi sembra una sorta di fallimento di quel sogno di "federazione degli Stati europei" che uno dei fondatori dell'Unione europea, l'italiano Spinelli, auspicò Pertanto, esprimo il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori - fortemente europeista come lo fu Spinelli - sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo. Chiedo

Lo Staff College è nato come programma speciale delle Nazioni Unite nel 1996 e, con deliberazione dell'Assemblea generale, tale istituto è diventato agenzia autonoma, con sede a Torino, in un un *campus* dedicato ad attività internazionali di non grandi dimensioni, ma di grande significato. Credo che esso costituisca un piccolo gioiello della città di Torino.

lo Staff College*,* che ha come missione la formazione di funzionari internazionali nell'ambito della famiglia delle Nazioni Unite, anche con l'ambizione di infondere un po' di spirito manageriale, che aiuti nella gestione delle complesse attività delle Nazioni Unite, soprattutto nell'ambito dello sviluppo economico, della cooperazione, della pace e della sicurezza.

chiarisce quali sono le prerogative di questa piccola istituzione: l'autonomia e l'immunità dei funzionari, l'inviolabilità della sede, l'esenzione dalle imposte italiane dei funzionari, ed analoghe disposizioni. Ripeto, è una piccola ma importante realtà: lo Staff College*,* insieme alle altre due agenzie, occupa un *campus* moderno

e l'ONU sullo *status* dello Staff College del sistema ONU in Italia è infatti di indubbia utilità. Ricordo che lo Staff College nasceva nel 1996 come programma quinquennale affidato al centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), con sede a Torino, e che dal 1º gennaio 2002 divenne un organismo autonomo...

Ricordo che lo Staff College nasceva nel 1996 come programma quinquennale affidato al centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), con sede a Torino, e che dal 1º gennaio 2002 divenne un organismo un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio dotato di un proprio statuto che ne regola il funzionamento; esso opera sulla base di determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguardanti principalmente i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace, della sicurezza e della gestione interna del sistema delle Nazioni Unite. È stata inoltre sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali, campo in cui lo Staff College rappresenta un riferimento di eccellenza nel settore della formazione manageriale. Fatta questa breve, ma doverosa premessa e sorvolando su un puntuale commento del testo dell'Accordo di cui si discute oggi, occorre dire che esso riguarda degli aspetti funzionali dell'organismo, che mi eviterò ed eviterò ai colleghi di passare in rassegna, visto il disinteresse che stanno dimostrando per questi argomenti internazionali. Non vorrei ripetere quello che ho detto giovedì, ma quasi mi si costringe Vorrei solamente porre l'accento, così come ha fatto il collega Evangelisti nell'altro ramo del Parlamento, sul fatto che lo Staff College è un'istituzione, Vorrei solamente porre l'accento, così come ha fatto il collega Evangelisti nell'altro ramo del Parlamento, sul fatto che lo Staff College è un'istituzione, peraltro voluta dall'allora segretario generale dell'ONU Boutros-Ghali, destinata a fornire uno strumento completo ed efficace di apprendimento per il sistema ONU, e quindi a rafforzare la capacità dello *staff* ONU di raggiungere importanti obiettivi di cambiamento e di realizzare appunto concretamente ed efficacemente gli obiettivi che l'ONU stessa si pone. inutile continuare ad argomentare, poi, sull'indubbia utilità della realizzazione di detto progetto con riguardo alla localizzazione di tale organismo.

per la proroga degli interventi di cooperazione, sviluppo e sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

mentre normalmente questo tipo di materia viene regolato con un disegno di legge ordinario di iniziativa parlamentare. Il decreto-legge in esame finanzia o prolunga il finanziamento delle missioni italiane all'estero fino alla fine del corrente anno, per due mesi.

che contribuiscono alla ricostruzione, alla stabilizzazione e al sostegno dei processi di pace nei Paesi in cui il nostro Governo e le nostre Forze armate sono intervenute.

In Afghanistan la nostra azione è volta a portare a termine gli impegni previsti, con l'assegnazione di un contributo volontario verso il *Civilian Surge,* con particolare riferimento all'area di Herat. Abbiamo poi altri interventi, sempre nella medesima area, di cui sottolineo solo il *World Food Programme* per la sicurezza alimentare delle popolazioni civili afgane presenti in questo territorio.

Inoltre l'Italia continua a favorire la ricostruzione, mediante taluni finanziamenti, in alcune zone particolarmente fragili e bisognose del nostro intervento.

dove si continua ad operare tramite gli organismi internazionali. Quanto al rapporto con gli organismi internazionali, sottolineo che il nostro impegno è destinato a contribuire

un attimo - c'è la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.

operazioni di polizia significative, come quelle della Guardia di finanza, che esercita un'attività di controllo in Libia, in Afghanistan, in Kosovo, Allo stesso modo, per i Carabinieri vi sono grossi impegni, in termini addestrativi soprattutto, per le forze di polizia in Iraq e in Afghanistan. Altri aspetti interessanti delle nostre missioni sono rappresentati dall'attività addestrativa che le nostre forze svolgono nei confronti delle Forze armate (non di polizia) sempre in ambito di Afghanistan e Iraq. attività sono particolarmente significative, perché a loro fa riferimento quella discussione continua del fino a quando rimanere in Iraq e in Afghanistan: la soluzione che si delinea o che si adombra è sempre quella di avere la possibilità che alle forze delle Nazioni Unite presenti per svolgere le operazioni di pace si sostituiscano progressivamente, in termini operativi e in termini di responsabilità, le forze di polizia e le Forze armate di questi due nuovi Paesi. Un grosso impegno per il loro addestramento è svolto dalle Forze armate e dalle forze di polizia italiane.

del contratto sottoscritto con lo Stato i volontari che, impegnati in missioni internazionali, vedano scadere il periodo per il quale avevano confermato il loro dovere, e che possa essere richiamato per esigenze

che riguardano la doverosità di risarcire il personale che ha subito danni, presumibilmente da radiazioni di uranio impoverito;

la liquidazione di materiali, il cui rimpatrio non è più conveniente, a favore dei Paesi nei quali questo materiale è stato impiegato. Il decreto contiene poi disposizioni che riguardano la del trattamento per il personale civile che partecipa alle operazioni di pace a quello previsto per i militari; vi è una disposizione particolare sull'allungamento della permanenza in attività degli organi di rappresentanza, la cui scadenza del mandato sarebbe i primi dell'anno 2010 e che viene invece procrastinata dal

per il 2009 era prevista una copertura finanziaria di un miliardo di euro; sommando però le coperture dei sei mesi più i quattro mesi più gli ultimi due mesi attuali, siamo giunti ad un miliardo e mezzo di euro, il che vuol dire che non è vero che nel momento in cui si deve stabilire una copertura si mette in discussione la possibilità di effettuare

finanziaria per il 2009, relativamente alle somme appostate per il bilancio del Ministero della difesa a condizione che fossero integrate con 500 milioni

Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, è stato detto da molti, ed io concordo, come l'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisca un aspetto importante dell'azione internazionale del Paese ed un elemento essenziale e qualificante della nostra politica estera e di difesa.

si riesce a mantenere un livello di inquinamento acustico accettabile per consentire agli oratori di intervenire. Si può ben dire che questo sostegno e questa fiducia siano stati innanzitutto merito dei nostri militari impegnati nelle missioni internazionali. È infatti risaputo com'essi siano tra i più apprezzati in questo tipo di lavoro: e non perché assistono i bambini (si è fatta anche della facile ironia su questo da parte di qualche nostro alleato). A ben vedere, si tratta anche di questo, cioè del fatto che una missione di pace non può non comportare una dimensione anche umana. La verità è che i nostri militari sono apprezzati per il fatto che sanno combinare l'efficienza militare con una grande capacità politica. Sono del tutto condivisibili le parole di chi ha detto che creare la pace non è soltanto il compito di chi fa la sentinella contro i violenti, ma è anche il compito di chi sa disarmare gli animi e preparare le persone alla cultura della pace. È in ragione di tutto ciò che anche in questa occasione non mancherà il nostro voto favorevole alla proroga delle missioni internazionali delle nostre Forze armate e di polizia. È nostra convinzione, però, che questo passaggio parlamentare di rifinanziamento del nostro impegno internazionale non debba essere ridotto a *routine* ma debba e possa essere l'occasione per un confronto tra Governo e Parlamento sui temi della difesa e della e della politica estera. E allora voglio qui brevemente ricordare alcune criticità. La prima questione riguarda proprio l'aspetto finanziario. Nel merito del provvedimento, osserviamo che, con riferimento all'assetto globale delle nostre missioni, il decreto opera alcune scelte. In particolare, confrontando le risorse stanziate per le tre missioni principali, si rileva quanto segue: la missione ISAF dispone per il bimestre in corso di 22 milioni di euro in meno rispetto al bimestre precedente; la missione UNIFIL (Libano) dispone sempre per il bimestre in corso di 10 milioni di euro in meno; infine, le missioni nei Balcani dispongono per il bimestre in corso di 6 milioni di euro in meno. Gli stanziamenti ridotti preludono ad un ridimensionamento dei contingenti che operano nei Balcani e in Libano. Anche in questo caso l'eventuale riduzione dovrebbe essere dettata da valutazioni politiche sottoposte alla discussione parlamentare e dall'andamento del conflitto in atto in quelle aree e non da esigenze puramente contabili. Quanto al disimpegno dei nostri contingenti dai Balcani, ed in particolare dal Kosovo, vi ricordo che quell'area continua ad essere interessata da una situazione di conflitto latente, specie nella Bosnia-Erzegovina e nel Kosovo. Pertanto una riduzione del contingente potrebbe avere effetti seriamente negativi della stabilità dell'area. In Kosovo ci sono segnali particolarmente preoccupanti. Il 15 novembre si sono svolte le prime elezioni politiche e municipali dopo la dichiarazione di indipendenza del 28 febbraio 2008. Le elezioni si sono svolte in modo sostanzialmente pacifico, anche se Belgrado ha invitato la comunità serba al boicottaggio. Ma negli ultimi giorni si è registrato un grave attentato. Soprattutto, il 24 novembre la Serbia ha realizzato una nuova base militare a ridosso del confine con il Kosovo. La maggioranza albanese che vive nella zona ha espresso la propria insoddisfazione per la decisione di Belgrado, giudicando la mossa come una dimostrazione tesa ad intimidire la popolazione. Insomma, l'Italia, che evidentemente ha più interesse di altri Paesi alla stabilità dell'area, deve seguire la situazione con particolare attenzione ed eventuali riduzioni delle truppe devono essere ben valutate. Colleghi, il Senato ha approvato pochi giorni fa una manovra finanziaria che cancella il finanziamento del fondo per le missioni internazionali per il 2010. Vale a dire che, mentre dal 2003/2004 tutti i Governi che si sono succeduti hanno agito per assicurare una dotazione finanziaria strutturale all'impegno italiano nelle missioni di pace, dal prossimo 1° gennaio si dovranno di volta in volta andare a cercare le risorse necessarie nel capitolo delle spese impreviste. Scelte strategiche per il Paese, che dovrebbero competere esclusivamente al Ministero della difesa e al Ministero degli affari esteri, nel quadro di una politica complessiva, saranno dettate, non da valutazioni politiche, ma da decisioni di cassa. Una situazione cui bisognerà porre rimedio se non si vorrà gettare sui nostri militari impegnati nei diversi teatri operativi il peso dell'incertezza e della provvisorietà della politica che la soluzione trovata con la presentazione dell'emendamento depositato questa notte alla Camera, che rimette la copertura delle missioni militari di pace a risorse derivanti dallo scudo fiscale, non ci sembra adeguata. L'emendamento definisce infatti anche il procedimento con cui queste risorse saranno rese esigibili. Tale procedimento prevede una ripartizione tra molti Ministeri destinatari di queste risorse, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimeranno il parere

sia per i nostri militari che per tutta l'opinione pubblica nazionale. Infatti, va detto con forza che tener conto delle disponibilità finanziarie, attuando ogni evidente razionalizzazione possibile, non significa assolutamente privilegiare profili di politica economica rispetto a problematiche di politica estera.

a finanziamenti per le missioni per un bimestre, come in questo caso, è stato scelto correttamente, in quanto si era intravista una possibilità di rimozione progressiva degli impegni. Va ricordato quindi che questa limitata durata dell'intervento di rifinanziamento risponde all'esigenza, anzi all'opportunità, di intervenire con tempestività rispetto al mutare degli scenari di impegno dei militari nei diversi Paesi interessati. quindi condivisibile il comportamento del Governo, che ha optato per una proroga più corta, in coincidenza anche dell'eccezionale congiuntura economico-finanziaria, con la la speranza di poter ridurre la consistenza di alcuni interventi. Si ritenevano infatti possibili in particolare una contrazione degli impegni in Afghanistan, in conseguenza della fine del processo elettorale, che sarebbe culminato nel voto del 20 agosto, ed eventualmente anche una rimodulazione degli interventi dei Balcani e in Libano.

risulta coerente con quanto dichiarato in queste ore anche dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ossia che, attraverso un ulteriore sforzo in terra afgana, che ha quale finalità una precisa ed esplicita *exit strategy*, andiamo però a calendarizzare un futuro più razionale per un disimpegno. Si tratta quindi di un disimpegno progressivo, fissato in precise scadenze, man mano che gli afgani prenderanno democraticamente il controllo del loro territorio. L'altro punto forte della nostra strategia sarà anche il rilancio della collaborazione con il Pakistan tra i vari e numerosi obiettivi delle nostre missioni internazionali, non possiamo comunque dimenticare - anche perché si sta intensificando - la caccia necessaria ai signori della droga *made in* Afghanistan. Nella lista dei talebani pericolosi compaiono 50 nuovi nomi, legati proprio alla lotta ai trafficanti di droga.

sintonia con gli alleati, e in particolare con quello americano, anche il nostro Governo si aspetta dal nuovo Governo afgano e dal Pakistan, anche in cambio degli aiuti attuali e prossimi futuri, impegni precisi nella lotta al terrorismo e alla criminalità,

Il prestigio ed il ruolo vitale nel nostro Paese nella politica estera e di difesa si palesa anche fra la nostra società civile. Infatti, il nostro Governo, le istituzioni ed il Paese tutto vogliono dimostrare con ogni mezzo la ferma vicinanza ai nostri uomini impegnati nelle varie missioni internazionali. vi è stata la recente istituzione di una giornata commemorativa per le vittime del vile attentato terroristico del 12 novembre 2003 a Nassiriya. Inoltre, vorrei poter menzionare il fatto che lo scorso 14 novembre, presso un Comune in Provincia della mia Vicenza,

l'impegno dell'Italia è quello di fornire un contributo costruttivo all'edificazione di un sistema internazionale sempre più efficiente, quale risposta appropriata alla complessità delle sfide e delle minacce che la comunità internazionale deve affrontare quotidianamente: dai conflitti armati più o meno estesi, al terrorismo, dal traffico di esseri umani, di armi e di droghe, alla pirateria in mare. Un impegno importante in termini di risorse umane e finanziarie. L'Italia, come parte dell'Unione europea, della NATO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'OSCE, è ormai inserita in attività operative internazionali di varia natura, in un *team* globale e cooperativo di risposta alle specificità delle crisi. Ciascuna delle attività operative a cui partecipa il nostro Paese in ambito internazionale ha come unico obiettivo quello di proteggere la popolazione civile, favorire i processi di pace e di stabilizzazione interna nella fase di transizione. azioni che, viste unitariamente, si avvalgono del dialogo diplomatico, della presenza militare, di interventi di varia natura volti a favorire una ricostruzione del tessuto socio-economico dell'area interessata, attraverso l'approvazione di programmi nazionali di cooperazione bilaterali e multilaterali. Le missioni militari internazionali, per come sono pensate ed autorizzate, promuovono quindi ciò che è contenuto nei principi generali enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani: sedano quegli atti che per la loro gravità, disconoscendo e disprezzando i diritti dell'uomo, possono giungere a destabilizzare o a mettere in pericolo la libertà, la pace e la sicurezza nel mondo. Noi europei abbiamo ribadito questo impegno di visione alta dell'umanità, pacifica, libera, operosa, unita da relazioni amichevoli, quando abbiamo deciso di redigere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, confluita poi, nel 2004, nel Trattato di Costituzione europea. Per tali ragioni, la presenza di militari italiani all'estero è un atto necessario di *partnership* internazionale, che viene posto in esecuzione solamente quando una situazione specifica degenera in scontro interno, generando conseguentemente problematicità e ripercussioni esterne, tanto da non poter essere più ignorata. ignorata. In quel momento, allora, la presenza fisica di Stati coesi e solidali in una determinata area diventa la modalità di superamento dei conflitti e di protezione e salvaguardia della vita e di interessi collettivi. È sicuramente una scelta non facile, ma è una scelta politica ineludibile, se vogliamo che alla comunità internazionale vengano garantite pace e stabilità e che le tensioni possano essere solamente dei momenti isolati, contenuti e brevi, di crisi interna, nei quali la comunità internazionale non si porge come frammentata, debole e vulnerabile, ma come un soggetto che, posto innanzi a situazioni di pericolo, reagisce in modo corale, condividendo con determinazione scelte strategiche, azioni e obiettivi finali. L'assenso che il Governo e il Parlamento danno alle missioni internazionali scaturisce da una decisione cosciente e ponderata, forte della certezza che ciò servirà in qualche modo a rendere l'area d'intervento più stabile e sicura. Il Governo e il Parlamento debbono vigilare affinché le amministrazioni della Difesa pongano costantemente in essere, con la flessibilità che la situazione ed i contesti richiedono, tutte le misure di sicurezza, di addestramento, di informazione necessarie a proteggere la vita dei nostri soldati, nella volontà di evitare la benché minima possibilità di errore nelle operazioni e di ulteriori lutti.

del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base della rappresentanza delle Forze armate, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. La relazione illustrativa al provvedimento specifica che l'urgenza dell'intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo dei suddetti organi deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato in corso. La decisione del Governo di prolungare il mandato di organismi a carattere elettivo è un atto che in noi desta perplessità: in primo luogo, perché viene inserito in un provvedimento riguardante le missioni internazionali; in secondo luogo, per il fatto che tale proroga determina, in un periodo molto delicato nella vita delle nostre Forze armate, una frattura nel rapporto tra eletti ed elettori, i quali, come è noto, conferiscono legittimità a questi organismi di rappresentanza. Si palesa quindi il rischio di una possibile delegittimazione di tali organismi. È una preoccupazione che noi avvertiamo e che intendiamo sollevare in questa discussione, ritenendo che anche il Governo e gli stessi organi della rappresentanza militare la possano condividere. Proprio a evitare questo rischio, l'ordine del giorno G104 intende far sì che la proroga del mandato dei COCER permetta un effettivo rafforzamento del potere rappresentativo di tali organi, nel quadro del confronto iniziato in Commissione difesa sui vari disegni di legge di riforma della rappresentanza militare. È necessario, a nostro avviso, utilizzare proficuamente questa proroga, riempiendola di contenuti, soprattutto sul versante del rapporto fra l'attività dei COCER e le linee d'azione del Governo. A ben vedere, spesso e volentieri l'attuale Governo si è distinto nel non riservare l'adeguato ascolto nei confronti delle istanze provenienti dal mondo della rappresentanza militare. A tale proposito, si rammenta che, fatta eccezione per i 100 milioni destinati al comparto per valorizzarne la specificità, le richieste dei COCER sulla finanziaria sono rimaste, in realtà, quasi del tutto inascoltate. In particolare, per quanto attiene alla situazione contrattuale, va segnalato il fatto che si deve ancora giungere alla chiusura del biennio contrattuale 2008-2009, per il quale, fortunatamente, sono a disposizione risorse stanziate a suo tempo dal Governo Prodi. A rendere ancora più problematica la situazione si aggiunge la stessa riforma del modello contrattuale, che riserva al Governo la possibilità di erogare l'80 per cento degli aumenti contrattuali con decisione unilaterale, rimettendo agli esiti della contrattazione la sola quota residuale. Tutto ciò palesa il fatto che le richieste economiche contenute nelle piattaforme dei COCER e delle stesse forze di polizia ad ordinamento civile e militare andranno probabilmente deluse. Le cose non vanno meglio neppure in altri ambiti, signora Presidente. Ad esempio, il COCER chiede da tempo garanzie e soluzioni per evitare i tagli sul reclutamento, tagli che comportano il rischio di licenziamento per centinaia di volontari in ferma breve, che hanno già prestato servizio per 6-7 anni. Aggiungo finora, perché risulta che nel maxiemendamento alla finanziaria presentato alla Camera siano stanziate risorse per togliere il blocco del *turn over* per le forze di polizia. Questo alleggerirebbe, certo, la situazione anche per il personale delle Forze armate, sempre che venga confermata la riserva dei posti nei relativi concorsi ai volontari, cosa che dalla lettura del maxiemendamento non appare del tutto chiara. Anche in merito al piano alloggi, signora Presidente, il parere del COCER è, nei fatti, rimasto inascoltato. In conclusione, il ruolo degli organi di rappresentanza militare sostanzialmente compresso dalle decisioni governative e suscitano perplessità anche nella stessa base militare. Questa situazione, a nostro avviso, va assolutamente superata. Il Governo deve, nei fatti, riconoscere agli organi di rappresentanza la possibilità di essere valido e ascoltato interlocutore sociale per le materie di competenza. Questo è il senso del nostro ordine del giorno. *(Applausi senatore Di Giovan Paolo. o tecnico-organizzative. L'Italia è l'ottavo Paese fornitore di truppe all'ONU e il primo Paese in questo ambito dell'Unione europea. È mai possibile pensare di trattare questi argomenti senza discutere di politica estera

Mi pare che il nostro Governo, adagiato sulla certezza che, ovviamente, le nostre ragazze ed i nostri ragazzi vanno supportati, nutriti e protetti, non si ponga il problema di come le 33 missioni in 21 Paesi ed in due aree geografiche nascano o debbano finire, e perché, e di quanto incida sulla protezione delle missioni militari la spesa - o la non spesa, dovremmo dire - per la cooperazione internazionale e l'impegno del Ministero degli affari esteri nel mondo, praticamente semiazzerato. lo dico soprattutto ai colleghi relatori che ho apprezzato, e al Sottosegretario presente - vogliamo essere alternativi ma anche costruttivi. Con alcuni colleghi abbiamo non solo firmato l'ottimo disegno di legge della collega Pinotti, che dà un quadro alle missioni internazionali, ma anche proposto un disegno di legge costituzionale sugli articoli 78 e 79 della Costituzione che riprende la corretta riflessione fatta, da da posizione diversa, dal collega Ramponi: dobbiamo dare nella Costituzione una copertura alle nostre missioni internazionali all'estero e dobbiamo darla, secondo me, rispetto ad un quadro obbligatorio di legame con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Abbiamo poi presentato un disegno di legge per attribuire, caro Sottosegretario, ogni anno, nell'ambito della relazione del Ministro della difesa, truppe militari alle Nazioni Unite ed all'Unione europea: truppe alle Nazioni Unite per attuare lo Statuto delle Nazioni Unite e quindi permetterci anche di essere presenti nel Consiglio di Sicurezza quando vengono utilizzate le nostre truppe;

Questo è il nostro modo di essere costruttivi ed alternativi, cioè difendendo le posizioni per cui permettiamo ai nostri militari all'estero di fare il loro dovere

Un Governo ha il dovere di ricordare le vittime, di onorare i caduti, ma anche di fare fatti nuovi che consentano al Paese di avere delle leggi che permettano di operare.

La prima è che - a mio avviso - la situazione nella regione, in Afghanistan ma non solo, è molto più ipotecata per non dire più pericolosa

scorrendo le minute di tante riunioni dei Ministri degli esteri, non ho visto traccia di discussioni del genere. Certo, questa sera il Presidente degli Stati Uniti informerà

il rilancio civile, non c'è stata nessuna elaborazione europea e nessun Paese membro, neanche il nostro, si è fatto carico di dare questa priorità di elaborazione rispetto

senza un approccio regionale e senza chiamare a contribuzione e a responsabilità i paesi circostanti, ivi compresa la Cina, la mia profondissima convinzione, e non da oggi, è che non ci sia alcun verso di stabilizzare l'Afghanistan dall'interno.

ma non se ne verrà fuori senza prevedere una dimensione diplomatica regionale, con tutti i costi che ne derivano. La seconda questione attiene ad un tema che, immagino per tabù anche ideologico, non si vuole mai affrontare.

non dalla produzione di oppio, che potrebbe essere comprato, ridotto a morfina, con delle quote, come accade per la Turchia, l'Australia o la Spagna e altri Paesi

di narcotrafficanti, signori della guerra ed anche amministratori di grande rilievo, con una potenza e una capacità di corruzione delle istituzioni afgane che non saranno le nostre formazioni di 10, 15, 20 o 30 poliziotti in più ad arginare. So perfettamente che la comunità internazionale ha come una barriera ideologica a rispondere a questi problemi, ma il mio invito, da quando ho vissuto per sei mesi in Afghanistan, è volto a superare tale barriera. grazie al nostro proibizionismo gli afgani sono seduti su una montagna d'oro: è come se dicessimo agli arabi di non estrarre petrolio. petrolio. Possibile che non si possa almeno ragionare su come limitare i danni? E in un Paese seduto sopra la morfina la stragrande maggioranza degli ospedali opera senza anestesia, perché non c'è morfina.

mi piacerebbe pensare che con la forza delle nostre istituzioni saremo in grado di svolgere, prima della Conferenza del 28 gennaio, un dibattito con tutti i crismi in quest'Aula del Parlamento e mi piacerebbe che destra e sinistra, opposizione o maggioranza, si impegnassero in tal senso. Ci avviamo ad una presenza in Afghanistan di grandissima responsabilità e grandissimo rischio: lo dobbiamo fare sarebbe utile farlo in modo consapevole, per noi, per l'opinione pubblica e per i cittadini italiani.

è fin dal secondo dopoguerra che l'Italia partecipa a importanti missioni a carattere multinazionale che portano le sue Forze armate a prestare servizio fuori dai confini del Paese. L'Italia dei Valori riconosce pienamente l'importanza della partecipazione dell'Italia a dette missioni: siamo, infatti, convinti che non si possa prescindere da esse se si vuole perseguire una politica concreta di cooperazione in materia di affari esteri, difesa e più in generale di sicurezza per il nostro Paese. Non v'è, quindi, alcun dubbio che le Forze armate italiane rappresentino un elemento indispensabile per consentire al nostro Paese di assumere i propri impegni nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui è membro ed a cui far fronte con coerenza e successo.

e le loro missioni le più risolutive, ma anche le più sicure possibili. Proprio sulla base di tali convinzioni riteniamo che il metodo della decretazione semestrale, per consentire la proroga della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, non possa garantire al massimo livello la sicurezza di tutti i nostri operatori; figuriamoci quindi quella bimestrale come avviene stavolta. Proponiamo piuttosto una vera e propria riforma delle missioni, che possa assicurare il loro carattere pacifico e la sicurezza dei militari, obiettivi da perseguire tramite discussioni multilaterali da svolgersi nell'ambito degli organismi internazionali ONU e NATO. Se la cooperazione allo sviluppo cui l'Italia partecipa prevede un intervento pluriennale, l'Italia dei Valori si domanda come tale sviluppo possa essere raggiunto in soli 60 giorni. A tal riguardo, il mio Gruppo si era premurato di presentare nelle Commissioni 3a e 4a riunite degli emendamenti utili a prolungare il termine della copertura finanziaria fino al 30 giugno 2010. Chiediamo che in futuro si proceda con una legge di finanziamento che preveda una copertura economica triennale; ciò per consentire che l'intervento militare possa svolgersi in condizioni più tranquille e più sicure, soprattutto in quelle parti del mondo dove portare materialmente il nostro aiuto rappresenta un pericolo per i nostri stessi militari. signor Presidente e colleghi, in relazione al contenuto proprio di questo decreto, rappresento la contrarietà dell'Italia dei Valori al metodo con cui si pensa di far fronte agli impegni internazionali. Vi ricordo, colleghi, che parliamo di vite umane, di quelle dei nostri soldati e, una volta messe in sicurezza le loro, anche, ma non meno importanti, delle vite da salvaguardare di tutte quelle persone cui contribuiscono il *peace-keeping* e il *peace-enforcing* messi in atto dal nostro Paese. Giungo a trattare della dir poco delicata situazione dell'Afghanistan, dove riteniamo sia ormai difficile parlare di missione di pace, essendo quella regione un vero e proprio teatro di guerra, in cui l'Italia impegna il maggior numero dei suoi soldati. Non potrete certo negare che nello scenario afgano il numero di vittime, le modalità dello scontro e le dimensioni dei contingenti militari impiegati conducano a ravvisare una vera e propria guerra. Bisognerà ammettere che negli ultimi otto anni, da quando cioè ha avuto inizio la missione in Afghanistan, non si è raggiunto l'obiettivo di costituire istituzioni solide, in grado di dare sicurezza, stabilità e democrazia al popolo afgano. Probabilmente però questo fallimento non è imputabile alla quantità di uomini e strumenti militari impiegati, quanto piuttosto all'inadeguato sfruttamento delle capacità politiche, economiche e diplomatiche della comunità internazionale tutta. A questo punto, l'Italia dei Valori pretende di comprendere la linea che il Governo intende seguire in relazione a questa importante missione che ci vede coinvolti. Esprimiamo l'esigenza di una ridefinizione dell'intervento militare dell'Italia in Afghanistan, degli esiti di tale intervento militare e delle regole d'ingaggio. Richiesta, questa nostra, che si pone nella prospettiva di un progressivo disimpegno dei nostri ragazzi dalla regione, coerentemente con una *exit strategy* già sollecitata dal mio Gruppo. Per quanto non si possa nascondere il nostro imbarazzo nel rilevare il dietro front del presidente Obama - il quale, pochi mesi fa, aveva dichiarato di voler procedere al graduale ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, parole che si è poi rimangiato con la più recente decisione di inviare nuovi contingenti ciò non toglie, colleghi, che l'Italia non può sentenziare sul destino delle nostre missioni sulla sola base dei rapporti personali tra il nostro Presidente del Consiglio di turno e il Presidente degli Stati Uniti, per quanto quest'ultimo possa essere un eccellente rappresentante democratico e l'ultimo premio Nobel per la pace. Ricorderete tutti, colleghi, cosa fu scritto all'articolo 11 della nostra Costituzione nel 1946. Non è forse vero, dunque, che l'Italia sa sfruttare meglio i suoi mezzi politici, economici e diplomatici di quanto non sappia fare con la guerra? Dovrebbe ricorrere di più a certi strumenti per mantenere alto il suo impegno internazionale. Questo ormai consolidato modo di procedere non fa che defraudare, in maniera sempre più preoccupante, il nostro Parlamento del suo ruolo specifico. E l'Italia dei Valori non si stancherà mai di imputare a questo Governo l'arroganza di voler bypassare regolarmente la funzione e l'impegno per cui siamo chiamati qui a svolgere il nostro lavoro. Per quanto ci si possa ritenere soddisfatti che in questo decreto ci si sia ricordati di rifinanziare, anche se solo per due mesi, la cooperazione allo sviluppo il fondo per lo sminamento umanitario, che sono tutte cose degne di nota, è impensabile ed inaccettabile che non si sappia neppure come fare a programmare il nostro impegno all'estero dal 1° gennaio: non un solo euro è destinato nella finanziaria per i prossimi anni al fondo per le missioni internazionali, che i Governi di centrosinistra avevano previsto e finanziato all'articolo 1, comma 1240, della finanziaria per Inoltre, anche se meno importante, ma sicuramente esemplificativo della situazione delle nostre Forze armate, all'articolo 3, comma 7, si prevede la proroga per decreto, per ben due anni, della rappresentanza militare tutta. Mi auguro sia chiaro come, così facendo, si attenti al principio democratico della rappresentanza elettiva. La giustificazione presentata è che non si farebbe in tempo a svolgere le operazioni elettorali. Se così fosse, forse si potrebbe varare per decreto una modifica delle procedure così articolate, non la proroga di rappresentanti eletti ormai anni fa e che dovrebbero peraltro occuparsi di tenere le relazioni con l'amministrazione nella delicata fase del passaggio alle Forze armate professionalizzate. Inutile dire che non siamo d'accordo. Riteniamo semmai più opportuno pensare a una norma che provveda allo snellimento della procedura d'elezione anziché autorizzarne lo slittamento. Anche di questa improprietà abbiamo voluto discutere nelle relative Commissioni. Ciò che più di tutto il mio Gruppo auspica è che questo Parlamento non resti del tutto sordo alle perplessità espresse in più occasioni dall'Italia dei Valori. L'augurio è che tutti voi prendiate coscienza del fatto che la forma della decretazione semestrale o, peggio ancora, più breve, non è degna di regolare questioni delicate come quella della vita dei nostri ragazzi inviati all'estero. Continuiamo a nutrire la speranza che tutti prendano coscienza di quanta responsabilità ci è stata affidata e di quanto sia dovuto agli italiani, ossia un completo e serio dibattito parlamentare su temi come quelli trattati dal decreto-legge oggi in

n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»; e di polizia. Il dibattito nel merito dell'opportunità della presenza, e anche di molte delle questioni che sono state al centro di alcuni degli interventi che mi hanno preceduto,

della misura che ci viene sottoposta per il voto, ma soprattutto - ripeto - nella maggior parte degli emendamenti proposti dalla maggioranza,

Sottoscrivo in pieno, salvo la parte finale, l'intervento del senatore Pegorer e quindi le critiche puntuali che egli ha mosso in merito al comma 7 dell'articolo 3 del provvedimento che ci apprestiamo a votare, relativamente al congelamento del rinnovo degli organismi di

Oggi non parliamo delle missioni italiane all'estero. Non parliamo neanche del valore umano che caratterizza - unica nota positiva - la nostra politica internazionale, perché se dovessimo stare dietro alle frequentazioni del Presidente del Consiglio non ci sarebbe niente di cui essere felici. Oggi parliamo di un altro

coinvolti sul fronte delle difese interne, è la lotta al terrorismo internazionale. L'opinione pubblica a fatica,

non siamo in Afghanistan per problemi afgani, ma perché il terrorismo internazionale interessa tutte le democrazie occidentali più o meno colpite o minacciate da questo fenomeno. Allo stesso modo la nostra presenza

i nostri eserciti all'estero oggi servono proprio per garantire la sicurezza interna e la democrazia all'interno degli Stati. Premesso ciò, approfitto della presenza del sottosegretario Cossiga per rivolgere un invito al Governo.

fino alle basi afgane, internazionali, ONU e italiane. L'Emirato ha grande interesse a rapportarsi con l'Italia, oltre che con tutto il mondo occidentale.

allungare pertanto queste missioni di qualche ora per mantenere buoni rapporti con questo Emirato che tanto interesse, anche economico, ha nei nostri confronti.

Stiamo approvando un atto che sta diventando solito nella nostra azione parlamentare, ovvero il rinnovo delle missioni internazionali,

versare del sangue; è una missione su cui l'Italia da subito si è impegnata in modo molto significativo; eppure in questa discussione sembriamo soltanto in attesa di una strategia che deve essere disegnata altrove. Più volte in questo Parlamento abbiamo detto è importante che l'impegno militare sia l'elemento fondamentale per poi poter incidere nelle dinamiche di politica estera e in Italia, ancora prima che in molte altre Nazioni, abbiamo espresso l'esigenza che la missione in Afghanistan

Ebbene, ad agosto, per chi ha avuto la voglia di leggere i giornali in spiaggia o in montagna, si è aperto un dibattito, con una prima intervista del Ministro della difesa cui è seguita una serie di risposte, nelle quali si diceva (talvolta facendo un po' di confusione e mettendo insieme regole di ingaggio e codici militari, che sono due cose diverse) che la

l'azione propria delle missioni internazionali. Ebbene, penso sia importante impegnare il Governo perché quanto prima questo auspicio agostano riportato dalla stampa, che poi non ha avuto, purtroppo, un seguito settembrino nelle Commissioni parlamentari, approdi all'approvazione di un nuovo codice che contempli la fattispecie specifica di come oggi gestiamo la sicurezza con le Forze armate, che è quella delle missioni internazionali.

Il voto che si appresta a dare l'Aula sul provvedimento di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali è - come dichiarato da tutti - estremamente importante per il nostro Paese. Ci rende orgogliosi e partecipi del ruolo strategico che le nostre Forze armate svolgono a tutela di valori - dobbiamo ricordarli - universali e irrinunciabili, quali la pace e la democrazia. I nostri militari sono là per queste missioni specifiche. Il nostro Paese sta sostenendo uno sforzo imponente e costoso e quindi è molto difficile

Paesi. Ricordo che abbiamo una condotta contemporanea di circa 30 missioni in 20 differenti parti del mondo, per una presenza media superiore a 8.600 militari: dati ancora più rilevanti se rapportati alle perduranti difficoltà economiche mondiali, che rendono specialmente difficile, e dunque meritorio, il rispetto da parte dell'Italia degli impegni assunti in ambito internazionale. Non possiamo infatti dimenticare che la fine della Guerra fredda e la caduta del Muro di Berlino - di cui poche settimane fa abbiamo celebrato il ventennale hanno modificato indelebilmente lo scenario strategico mondiale e, con esso, il ruolo del nostro Paese e il ruolo delle sue Forze armate. Si è assistito ad una sostanziale diminuzione della presenza in Europa e nel Mediterraneo di forze militari ostili in grado di portare nel medio termine minacce dirette al territorio nazionale. Al contempo, da un lato, si sono moltiplicate nelle varie zone del mondo - Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Iran, Somalia - le crisi regionali

terroristica - di matrice prevalentemente islamica, concretamente in grado di elevare l'entità del pericolo a livelli in passato inimmaginabili. Di fronte a questa nuove sfide, l'intera comunità internazionale è chiamata a svolgere un ruolo attivo, perché il mantenimento della pace e della sicurezza non può essere appannaggio e e responsabilità di pochi, ma deve essere un dovere di tutti i Paesi democratici, prevalentemente ricchi e industrializzati, a sostegno delle democrazie più povere e in maturazione. L'Italia e le sue Forze armate hanno risposto con grande coraggio, senso del dovere, professionalità e capacità operative non comuni, facendo guadagnare al nostro Paese un significativo prestigio internazionale e un apprezzamento unanime nell'ambito di tutti i consessi mondiali ai quali ho partecipato e partecipano i miei colleghi.

in genere indifesa, povera e tristemente attanagliata da questi gravissimi problemi mondiali. Per questa via le missioni internazionali si sono rivelate uno strumento straordinario per tenere alto il nome dell'Italia all'estero, dove i nostri militari, ripeto, sono particolarmente apprezzati, perché sempre attenti a stabilire un contatto umano con le popolazioni locali. Prova ne è il recente elogio espresso dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nei confronti dell'Italia per il ruolo svolto in numerosi teatri di crisi, con particolare riguardo all'Afghanistan, cui è seguita la richiesta di un rafforzamento del nostro impegno, che mette in primo piano la ricostruzione del Paese, la crescita, l'efficienza dell'apparato amministrativo, l'assistenza, l'addestramento e, soprattutto, il sostegno alla popolazione civile. Come Parlamento attendiamo le proposte che il Governo formulerà su quello che potrà essere l'apporto dell'Italia alla nuova fase del processo di sviluppo e pacificazione dell'Afghanistan, convinti della grande responsabilità cui siamo chiamati e alla quale, ripeto, non possiamo sottrarci.

I nostri alleati devono sapere, senza se e senza ma, che la volontà politica dell'Italia rimane quella di continuare a contribuire con un impegno che,

Vi sono altri motivi per i quali la nostra azione in Afghanistan si sta conducendo in un certo modo.

quindi che è anche un nostro interesse nazionale difendere la sicurezza globale per non trovarci poi in questo ingranaggio. La seconda ragione per la quale il nostro impegno deve essere approfondito e conosciuto fino alla fine, è che in quella regione contribuiamo a promuovere la democrazia di tutti. Lo stiamo facendo dall'interno: ha ragione la presidente Bonino, non dobbiamo fare pressioni dall'esterno verso un Paese. Siamo convinti

l'Afghanistan si sta proponendo come un test che non può fallire. È un test per la credibilità della NATO, che per la prima volta si impegna con un'entità enorme di risorse fuori dall'area per la quale è competente. Inoltre, siamo di fronte ad un test per i rapporti transatlantici: questa missione ha messo in luce il rapporto chiave tra Europa e Stati Uniti, che non è mai stato così convinto convinto e profondo come in questo momento; giustamente, è anche stato ricordato che domani avremo la sensazione e la contezza degli impegni che gli Stati Uniti vogliono continuare a prendere in quel territorio. Si tratta però anche un test per i rapporti NATO‑Russia: per la prima volta la Russia collabora pienamente, concedendo i diritti di transito e di sorvolo, cosa che non aveva mai fatto.

credo che occorra un obiettivo preciso, che non può essere soltanto il fatto che l'Afghanistan si avvicini ad un modello di democrazia occidentale che sarebbe una forzatura - ma che sia un Paese autosostenibile. E qui vengo a quello che diceva la collega Bonino, per cui non possiamo trascurare l'impegno regionale, che dobbiamo invece favorire in questo territorio.

di sollevare quel territorio e quella Regione per farne, non già un'appendice del mondo occidentale, ma uno spazio di democrazia nel territorio in cui si opera. *(Applausi

Concordo con il senatore Di Giovan Paolo che, a sua volta, richiede questo benedetto dibattito e si rammarica perché in quest'Aula si parla di tutto meno che di quello, come afferma il senatore Perduca.

o la soluzione di situazioni contingenti riferite alla difesa e, molto spesso, riferite alle missioni. Vi prego di perdonarmi per l'emendamento a mia firma sul cambiamento del titolo,

induce, molto spesso, i parlamentari stessi ad approfittare di questo tipo di treno per risolvere problemi molto avvertiti dal personale e che giacciono per anni nelle Commissioni senza poter essere presi in considerazione.

Mi rimane da rispondere alla senatrice Pinotti che, appassionatamente, chiede l'approvazione di un disegno di legge che dia un contesto giuridico adeguato alla realtà

debbo anche dire che il Governo ha promesso (e sta mantenendo tale premessa) di predisporre un testo che non sia solo una modificazione del codice militare di pace o di guerra ma un codice *ad hoc*. voglio ricordare a tutti coloro che sollecitano, giustamente, la necessità di un dibattito sulle operazioni che l'ordine del giorno da me fatto approvare

situazione di generale condivisione su questo provvedimento e in particolare, al di là della natura del provvedimento, della generale condivisione da parte delle forze politiche sul ruolo del nostro Paese nelle missioni internazionali, in particolare sul ruolo delle Forze armate, io sono costretto - e si tratta di una *excusatio petita* - a rispondere in primo luogo al senatore Marcenaro. In un intervento sull'ordine dei lavori, quindi estraneo di fatto a questa discussione questa discussione generale, egli ha voluto sottolineare come problematica l'assenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Comprendo le motivazioni e il quadro

disamina di alcuni punti relativi alle principali missioni all'estero, per poi provare a fornire elementi aggiuntivi in relazione alle problematiche sollevate dagli intervenuti. l'Afghanistan: è la missione sicuramente più importante, su cui molti degli intervenuti hanno concentrato la loro attenzione. La situazione attuale, come è noto, prevede una presenza di militari italiani nell'ordine di 3.150 unità sino alla fine dell'anno. Mi rendo conto che la peculiarità di questo dibattito, su un un decreto-legge che si occupa del finanziamento per gli ultimi due mesi, fino alla chiusura dell'anno, per le motivazioni che sono state peraltro compiutamente illustrate anche da alcuni degli intervenuti - i senatori Alberto Filippi e Galioto - limita in un certo senso i nostri margini di manovra. È evidente che, più compiutamente nei prossimi giorni e nel corso dei dibattiti che precederanno l'adozione del nuovo decreto per il finanziamento, a partire dal prossimo anno, alcune informazioni aggiuntive potranno essere date al Parlamento e vi sarà sicuramente occasione di approfondire alcuni temi. È stato più volte citato - questo sì che è vero - che si tratta di una prima volta. In effetti non si non si era mai fatto un decreto per due mesi. Questa peculiarità è legata in parte anche all'esaurirsi di quel fondo, previsto in maniera innovativa nel 2008: il fondo per le missioni internazionali in questo Paese non è una norma. È stato un tentativo, che ha avuto una sua efficacia nel corso dell'ultimo paio d'anni, ma che, come ha detto il relatore Ramponi, ha dimostrato anche un suo limite, suo limite, cioè che il fondo previsto per un valore complessivo di un miliardo si è in corso d'anno esaurito ed ha costretto il Governo a reperire, all'interno delle risorse peraltro disponibili, nuovi finanziamenti. Faccio presente che da questo punto di vista non posso che rivendicare come particolarmente significativo che per la prima volta con l'ultimo decreto - con questo si va sulla stessa linea - sia stato assicurato il pieno finanziamento anche degli oneri di preparazione delle missioni. Com'è noto, la gran parte degli oneri delle missioni sono relativi ai costi per il personale e, solo in parte, a quelli per le attività di preparazione di preparazione e di immissione in teatro. Questo nuovo approccio, che permette la totale copertura dei costi delle missioni, ha portato ad un rapido esaurimento di quel fondo ed alla necessità di reperire, come ha detto il relatore Ramponi, circa 500 milioni per la copertura dei costi totali. Da questo punto di vista, è stato più volte sollevato come la non conferma dell'esistenza di un fondo per le missioni possa essere vista come una diminuzione dell'attenzione del Governo alle missioni. Ebbene, evidentemente non è così. La volontà del Governo di continuare a garantire la partecipazione

fuorviante perché, a seconda del periodo considerato, rischiano di essere incluse spese che per natura sono ripetitive di mese in mese con spese invece *una tantum*. Tornando comunque al dettaglio della situazione come è noto, è in corso una profonda rivisitazione degli obiettivi, non solo militari, di questa missione. Nel corso del recente incontro a livello NATO in Slovacchia, a Bratislava, il generale McChrystal ha aggiornato tutti i Ministri dell'alleanza sulla situazione e ha formulato una proposta per un nuovo approccio, approccio, tracciando peraltro una definizione delle necessità relative alle nuove risorse per attuare la strategia da lui proposta. Queste valutazioni, da un punto di vista generale, sono state ampiamente condivise all'epoca, anche se non ci si è ancora

le proposte di McChrystal sono attualmente al vaglio delle amministrazioni dei Paesi NATO. La senatrice Bonino ha voluto dare una visione forse eccessivamente Stati Uniti-centrica di ciò

quest'ultima che dovrà raggiungere una posizione comune. È evidente che, da questo punto di vista, sono in corso scambi

di eventualmente assicurare un suo contributo, cosa che non va vista come un semplice contributo di uomini aggiuntivi, ove necessario, ma come l'adesione ad una revisione di una strategia. Da questo punto di vista, sottolineo che quella che in sede NATO viene presentata come un *comprehensive approach*, cioè un nuovo approccio globale, non soltanto militare, alla situazione dell'Afghanistan, sia in effetti totalmente in linea con quella che è sempre stata la visione del Governo italiano su questa missione. Questo nuovo approccio si concretizza essenzialmente nell'adozione di quattro priorità fondamentali che sono state fatte proprie anche dal Governo italiano e sono alla base dell'azione politica del nostro Governo. è fondamentale mettere al centro dello sforzo collettivo della NATO, e quindi della missione ISAF, la popolazione afgana. Inoltre, è necessario accelerare ed intensificare ogni sforzo per sviluppare autonome capacità da parte delle forze di sicurezza afgane, ricercare un approccio più efficace, attraverso una maggiore sinergia tra l'attività dei vari partner internazionali, quindi agenzie civili nonché componenti militari,

in corso l'avvicendamento, ormai quasi completato, della Brigata Folgore, presente in questo teatro fino a poche settimane fa, con la Brigata Sassari. Contestualmente, come peraltro il Parlamento conosce, è stato programmato il rientro del contingente aggiuntivo che era stato inviato e si era trattenuto in Afghanistan durante il periodo elettorale. Questo per quanto riguarda le truppe sul terreno. Come già ho avuto modo di dire in Commissione, si sta anche completando la dislocazione in teatro di velivoli AMX, che sostituiranno i Tornado, nel quadro della caratterizzazione dell'intervento che è stata illustrata illustrata al Parlamento e che mira ad aumentare al massimo le capacità di ricognizione e di autotutela del nostro contingente. Per quanto riguarda il settore formativo e addestrativo delle forze di sicurezza afgane, come noto, la NATO ha avviato una nuova missione denominata «*NATO training mission-Afghanistan*», sulla falsariga di quella attualmente in atto in Iraq, che, a regime, dovrà consentire un maggiore coordinamento e una gestione unitaria delle attività addestrative cosiddette di *mentoring* delle forze di sicurezza delle forze di sicurezza afgane. Dopo l'Afghanistan vorrei passare brevemente ad alcuni punti relativi al teatro operativo libanese, che è stato citato dagli intervenuti. L'efficacia, e non la semplice presenza, della missione

Questo risultato è evidente ed è frutto del contributo decisivo della missione UNIFIL (che ha peraltro portato anche ad una forte credibilità delle Forze armate dell'esercito libanese), il che, com'è noto, non è merito di questo Governo, ma del Governo italiano. una missione fortemente voluta nella sua nuova configurazione dall'Italia e che l'Italia ha reso possibile in un momento estremamente delicato, al termine delle ostilità tra *hezbollah* ed Israele, promuovendo con l'invio di truppe la rigenerazione di una missione che era in corso da più di trent'anni e che aveva perso parte della sua efficacia. Da questo punto di vista, è noto l'apprezzamento per l'operato del nostro contingente; in particolare, va ricordata l'azione di comando del generale Graziano, il cui mandato, più volte rinnovato dal febbraio del 2007, volge ora al termine, anche a seguito della decisione dell'Italia di non presentare un candidato sostitutivo per permettere alla Spagna di poter

Da questo punto di vista, se è vero che attualmente le forze impegnate in teatro sono di poco superiori alle 2.100 unità, è evidente che, con il cambio del comando e con le diverse responsabilità di un Paese che non deve garantire il comando del contingente, la nostra presenza in questo teatro potrà diminuire, per contingente non superiore ai 400-500 uomini. Faccio presente, sempre nel teatro libanese, che nei prossimi giorni l'Italia assicurerà ancora una volta il comando della

In Kosovo, com'è noto, la mutata situazione sul terreno ha gettato ormai le basi per un passaggio della missione KFOR alla fase della cosiddetta *deterrence* *deterrence* *presence*, cosa che porterà ad un progressivo e graduale aggiustamento dell'impegno militare, nel senso di una diminuzione. Il decreto al nostro esame prevede sostanzialmente una presenza in Kosovo di poco superiore ai 1.900 uomini. coloro che sono intervenuti e che hanno fatto riferimento ad una volontà di disimpegno da parte del nostro Paese, dando una lettura di questo tipo ad alcune osservazioni avanzate recentemente anche

di procedere ad una riduzione unilaterale del proprio contingente: si arriva insieme e si va via insieme, quando le condizioni sul terreno lo permettono. Da questo punto di vista, come dicevo, la situazione in Kosovo è profondamente mutata. La NATO sta rivedendo della missione KFOR; soltanto all'interno di decisioni comuni potrà eventualmente essere rivista la presenza italiana. Com'è noto, è in corso di definizione una riduzione globale della missione KFOR in Kosovo, che nel corso dei primi mesi dell'anno prossimo potrà essere meglio definita. Si passerà così lentamente, nel corso dei primi sei mesi e quindi entro l'estate, ad una riduzione probabilmente probabilmente dell'ordine dei due terzi. Si tratta di aspetti che sono tuttora in discussione a livello NATO e che saranno sicuramente oggetto di ulteriore dibattito nelle prime settimane del prossimo anno. Per quanto riguarda la Bosnia, l'operazione Althea, guidata dall'Unione europea, in effetti ha ormai esaurito Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso pertanto di rimodulare la missione, attribuendole finalità puramente addestrative a favore delle Forze armate bosniache. Il nostro Paese ha avuto il comando di questa missione dal dicembre 2008, impiegando circa 270 militari. Questo permetterà una riduzione di circa 50 unità; non è molto, ma, come dicevo, soltanto quando sarà determinata una decisione comune da parte dell'Unione europea in relazione allo sviluppo nostro contingente. Un altro campo in cui siamo particolarmente impegnati, com'è noto, è quello delle operazioni antipirateria al largo del Corno

le tematiche che sono state sollevate dal senatore Di Giovan Paolo ed in parte anche dalla senatrice Bonino e dalla senatrice Pinotti, il Governo segue con grande interesse le attività parlamentari, in relazione anche alle modifiche del contesto costituzionale, che potranno portare in futuro ad un nuovo approccio nel rapporto tra Parlamento e Governo in relazione alle missioni. Tuttavia in questo momento non possiamo che continuare com'è ormai prassi consolidata: Un ultimo punto, cui ha fatto riferimento la senatrice Pinotti, è quello relativo all'evoluzione dei codici penali militari. Da questo punto di vista, sono terminati i lavori di un'apposita Commissione all'interno del Ministero della difesa e, della difesa e, a brevissimo, il Governo fornirà nuovo impulso all'attività (che è già nata in Parlamento) di creazione di un nuovo codice, più adatto alla tipologia di missioni che svolgiamo rispetto agli antichi codici penale militare di pace e penale militare di guerra,

sulla costituzione in giudizio del Senato in ordine a due conflitti di attribuzione. Le votazioni saranno effettuate nel corso della seduta antimeridiana in orario che la Presidenza comunicherà, previo accordo con i Capigruppo. **Sulla votazione

sia per fatto personale. Nella suddetta interrogazione, sottoscritta dall'intero Gruppo IdV del Senato, citando articoli di stampa che facevano riferimento al presidente della CONSOB Cardia, chiedevo di sapere se rispondesse al vero che l'avvocato Marco Cardia, figlio del presidente della CONSOB, a libro paga di Giampiero Fiorani, ex «furbetto del quartierino», con una consulenza di 220.000 euro l'anno, fosse stato inserito nel comitato dell'Immobiliare lombarda, azienda del gruppo Ligresti, vigilata dalla CONSOB. Chiedevo inoltre di sapere se rispondesse al vero che l'avvocato Cardia avesse trasferito la sua residenza ai Parioli in un elegante complesso di proprietà della controllata Fondiaria, sempre del gruppo Ligresti. Dal Ministro

per presunta manipolazione del mercato dei titoli Unicredit, un vero e proprio falso, come risulta dall'atto 10981/09 della procura di Roma, che ha iscritto sul registro degli indagati Cardia e i soci di Unicredit per abuso d'ufficio e calunnia. Veniamo alle date, signor Presidente. trasmissione «Report» manda in onda un servizio sui derivati Unicredit, appioppati ad enti locali ed imprese. Il 15 ottobre deposito un esposto di denuncia a 10 procure della Repubblica contro i comportamenti fraudolenti di Unicredit in merito ai derivati affibbiati ad enti locali ed imprese fatte fallire (ricordo, ad

punire i comportamenti fraudolenti dei banchieri che spacciano montagne di derivati avariati commisurate alle *stock option* che incassano (vorrei ricordare, di Goldman Sachs solo per gratifiche natalizie), e disseminano povertà e miseria per le moltitudini, ha sanzionato un rappresentante dei consumatori

Nessuna marcia indietro sulla decisione di fermare la produzione di auto a Termini Imerese: quella di una riconversione ad altre produzioni «è una scelta che ha una base razionale ed economica» e quindi «non può cambiare. Quello che invece può cambiare è l'impegno per uno sviluppo diverso». Queste sono parole dell'amministratore delegato della FIAT, dottor Marchionne. Quella di oggi con il ministro Scajola è stata una trattativa vergognosa: in 20 minuti hanno deciso

La FIAT ha acquisito Chrysler, ha inglobato Bertone e ha tentato di comprare OPEL, ma poi chiude lo con la possibilità, peraltro, di modificare la produzione non si sa bene in cosa. Forse ne farà un supermercato o venderà motori, non lo sappiamo. Abbiamo 20 giorni per saperlo.

fronte ad un accordo al ribasso e anche all'ambiguità del ministro Scajola. Nei giorni scorsi avevo chiesto che il Ministro venisse in Aula e avevo chiesto al Presidente della 10ª Commissione di sentire in Commissione l'amministratore delegato Marchionne.

erogazioni ed incentivi: organizzi accordi di programma, faccia le cose in maniera dignitosa e da subito, entro 20 giorni, organizzi l'incontro con i sindacati e con le amministrazioni locali. Oggi sia Marchionne locali. Oggi sia Marchionne che le televisioni pubbliche hanno detto che il Governo regionale precedente doveva garantire determinate risorse. in questo momento ha messo a disposizione 400 milioni di euro e altri 100 milioni di euro li metterà il Governo. Non si capisce per quale motivo bisogna obbedire al diktat dell'amministratore delegato e chiudere Termini Imerese: è una cosa ignobile e inaccettabile!

Presidente, sono contento che il senatore Garraffa sia intervenuto con tanta enfasi sulle vicende che interessano la vita dello stabilimento di Termini Imerese.

Nessuno può pensare di invocare, così come stanno facendo alcuni partiti, interventi che non sono previsti dalle norme, né nazionali né comunitarie.

per fare un contratto di programma sono tali che alla FIAT non interessano. Infatti, per prendere 100 milioni di euro di fondi pubblici la FIAT ne dovrebbe mettere 800: queste sono le condizioni per fare un contratto di programma con una grande impresa.

e che chiedano alla FIAT di ripagare il Mezzogiorno e la Sicilia per ciò che hanno preso negli ultimi trent'anni, perchè se facciamo i conti di quanto ha preso la FIAT in Sicilia, il risultato è indecoroso, signor Presidente. Allora, che il Governo

relativa alla motivazione con la quale, in sede di appello, il tribunale dei minori di Napoli ha voluto respingere l'istanza per la concessione di misure alternative presentata dall'avvocato della giovanissima ragazza rom che è stata prima accusata e poi condannata a tre anni e nove mesi di reclusione per aver tentato di rapire una bambina. Questa vicenda è stata all'origine dei fatti gravi di Ponticelli, quando, tre anni fa,

appartiene a quella cultura e a quella comunità, quindi non può essere rieducata, non può essere portata in una casa perché, inevitabilmente e nuovamente, sarebbe soggetta a recidiva per quanto riguarda il reato. Credo sia la prima volta che in Italia viene emessa una sentenza così chiaramente ispirata a pregiudizi di tipo xenofobo. È qualcosa di grave che, dunque, deve vedere una reazione del nostro Parlamento. Ho presentato al riguardo l'interrogazione 4-02351 al Ministro della giustizia

di questa ragazzina che, evidentemente e palesemente, si trovava in quel contesto forse per rubare, certo non per rapire una bambina, fatto che poi non è avvenuto. Credo che una ragazzina come questa meriterebbe misure alternative di rieducazione. Certamente non possiamo accettare una sentenza che è in odore di razzismo. PRESIDENTE. Senatrice Carloni, la Presidenza prende atto della sua richiesta. **Sul futuro